Do comunicazione all'Aula dei risultati della Conferenza dei Capigruppo. dei Capigruppo. La Conferenza, riunitasi questa mattina, ha approvato all'unanimità il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 10 maggio. Per questa settimana rimane confermato il calendario già definito, salvo ulteriori determinazioni che potranno essere assunte dalla Conferenza medesima, già convocata per domani mattina alle ore 8,30. La prossima settimana, a partire dal pomeriggio di martedì 8 maggio, il calendario prevede l'esame dei disegni di legge sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione e per l'istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali, nonché di ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione competente. Nella seduta antimeridiana di mercoledì 9 maggio saranno effettuate le votazioni nominali con procedimento elettronico su una proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari relativa alla negazione di concessione dell'autorizzazione a procedere per reati ministeriali. Dopo lo svolgimento delle predette votazioni elettroniche preliminari, i senatori potranno comunicare il proprio voto in modo palese, fino alle ore 19, ai senatori segretari che ne terranno nota in appositi verbali. Infine, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che il Senato non terrà seduta nella settimana precedente le elezioni amministrative del 27 maggio. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1449.

Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, il decreto-legge di cui oggi si chiede la conversione afferisce

Infatti, essendo stata modificata la legislazione in tema di composizione dei Consigli giudiziari e a seguito dell'istituzione del Consiglio direttivo della Cassazione, non si è avuto tempo - anche perché questa legge non è ancora in vigore, c'è stata la proroga - e non c'è il tempo materiale per predisporre la normativa relativa alle elezioni e quindi anche tutto il supporto elettorale.

necessario proprio per approntare questo supporto elettorale, nonché per far approvare la legislazione relativa. relativa. Dico questo anche per rispondere, quasi preventivamente, sia all'ordine del giorno che agli emendamenti presentati, che tendono ad una riduzione di questo termine. Espressa questa esigenza, chiedo che il

di approvare la legislazione relativa all'istituzione del Consiglio direttivo della Cassazione. Tra un anno si potrà così votare per i due organismi e, in raccordo con la modifica dell'ordinamento giudiziario, avere più tempo

Il relatore ha dichiarato che c'era bisogno di un anno per poter predisporre i regolamenti e le attività necessarie per procedere alle elezioni dei Consigli giudiziari, così come previsto dal decreto legislativo

messo in atto appositamente per far sì che il provvedimento non venisse attuato. Questa è la verità: l'anno lo avevate già, perché non l'avete utilizzato? È questa la domanda a cui dovrebbero rispondere il relatore Di Lello e il Governo. Tra l'altro, è curioso curioso anche il fatto che il ministro Mastella, in qualità di senatore, sia sempre presente perché, come sappiamo, la maggioranza ha bisogno di tutti i senatori per votare, mentre oggi che si parla di una questione importante che riguarda il Ministero della giustizia il Ministro non c'è, come non è mai presente in Commissione quando si tratta di parlare dell'ordinamento giudiziario. Ciò è ancora più curioso e paradossale visto che l'articolo 110 della Costituzione riserva al Ministro della giustizia non tanto la predisposizione dei codici, non tanto l'elaborazione di leggi attinenti al codice penale, ai codici di procedura e quant'altro, ma i servizi della giustizia. Dunque, se esiste un provvedimento principe che riguarda direttamente il Ministro concernente materie che riguardano l'ordinamento giudiziario: ebbene, quando si parla di questo il Ministro non viene. Con tutto il rispetto per il sottosegretario Scotti, io credo che sia assolutamente necessario che il Ministro sia presente quando si parla di questi temi.

che, ripeto, anche formalmente, è stato paracadutato direttamente dagli uffici giudiziari in questa sede, senza nemmeno passare per l'elezione voluta dal popolo. Io credo che questo sia un dato assolutamente inaccettabile non soltanto inaccettabile, ma anche incostituzionale perché è del tutto evidente che non vi è alcuna necessità e urgenza di questo provvedimento. Le cosiddette necessità e urgenza nascono dall'assoluta inerzia del Governo che non ha messo in atto ciò che doveva provocando non soltanto un *vulnus* alla Costituzione, ma anche agli accordi presi in quest'Aula nel settembre scorso, quando si era dichiarato di far andare avanti alcuni decreti legislativi, intervenendo soltanto su tre

anche questo provvedimento, non lo si mette in pratica e poi si pone in atto sempre la solita tattica (magari dovreste anche cambiarla un po' e tentare qualche innovazione),

che si propongono continuamente provvedimenti che sono semplicemente rinvii che non sono dettati da nessuna reale necessità e urgenza, ma semplicemente dalla volontà politica. Io credo che sia un sistema di legiferare

magari domani potremo parlare anche di tali questioni; forse è impegnato su altri problemi che lui ritiene più importanti. Comunque, è del tutto evidente che non vi è alcun necessità e urgenza in questo provvedimento.

in realtà, sottolinea il fatto che tale decreto rinvia il termine per l'elezione dei Consigli giudiziari al prossimo anno e, per la verità, non censura il fatto del rinvio in sé, se ho ben capito; infatti, sbaglierebbe se lo facesse perché la necessità e l'urgenza non la leggiamo nel rinvio all'anno prossimo ma nel fatto che si doveva entro il 1° aprile procedere alle operazioni elettorali. In realtà, il collega Castelli fa un processo alle intenzioni. Lamenta il fatto che si sia voluto rinviare il termine perché il Governo avrebbe avuto il doloso intento di impedire l'applicazione di una norma di legge. Vorrei rispondere che quando si guarda alla necessità e all'urgenza, alla rispondenza ai requisiti costituzionali per quanto riguarda la decretazione d'urgenza, tutto va valutato al momento: urgenza e necessità vanno viste qui ed ora. Non si fa il processo alle intenzioni. Non è costituzionalmente rilevante se si ritenga colpevole o doloso il ritardo del Governo. Non è costituzionalmente rilevante che ci fosse un intento, anch'esso magari doloso, di rendere una qualche norma inapplicabile. Vero o falso che fosse, potrebbe essere politicamente censurabile

Tuttavia, questo non è - come dicevo - costituzionalmente rilevante. I dati sono chiari e sono quelli che ha esposto il relatore. Avevamo un termine al 1° aprile per lo svolgimento delle operazioni elettorali dei Consigli giudiziari. La disciplina applicabile a questo fine in un disegno di legge che è in corso di discussione e di esame in sede parlamentare; la data scelta per la proroga del termine

sarebbe stato probabilmente censurabile perché avremmo avuto un provvedimento d'urgenza del Governo su un meccanismo elettorale che concerne un potere autonomo dello Stato, qual è indubbiamente la magistratura. Dunque, sembra nel complesso corretto e rispondente a criteri di ragionevole esperienza e di razionale definizione dei tempi per la decisione legislativa

Siamo di fronte ai «si dice» questo o quel motivo, per cui questo o quel Ministro avrebbe voluto questo o quel ritardo. Ma di sicuro, signor Presidente, non siamo di fronte a questioni che abbiano un un rilievo dal punto di vista costituzionale. Rimangono nell'ambito della valutazione politica - certamente legittima - che l'opposizione fa, ma non incidono sulla legittimità costituzionale dell'atto.

Signor Presidente, prestare attenzione, come lei molto spesso ci ricorda, non è obbligatorio, quindi i colleghi che magari hanno voglia di fare altre cose le possono fare tranquillamente altrove e non in Aula. non in Aula. Come tutti sappiamo, nella scorsa legislatura la legge 25 luglio 2005, n. 150, ha conferito al Governo la delega ad emanare uno o più decreti legislativi di riforma dell'ordinamento giudiziario. Sostanzialmente, l'articolo 1 della legge indicata prevedeva undici interventi specifici oggetto di delega. In questa nuova legislatura, la quindicesima, con il varo della legge 24 ottobre 2006, n. 248, il Parlamento è già intervenuto su tre decreti legislativi, modificando il n. 106 del 20 febbraio 2006, avente ad oggetto, come tutti sappiamo, l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, e modificando anche il n. 109 del 23 febbraio 2006, che invece ha ad oggetto la disciplina degli illeciti disciplinari sempre con la legge che ho citato, quella del 24 ottobre 2006, questo Parlamento, invece, ha sospeso l'efficacia fino al 31 luglio 2007 del decreto legislativo n. 160 del 5 aprile 2006, quello relativo alla disciplina dell'accesso in magistratura e occorre precisare, rispetto a tale ultimo provvedimento, che è già iniziata la discussione in Commissione del disegno di legge presentato dal Governo. Oggi, invece, all'interno di questo panorama che riguarda comunque la riforma dell'ordinamento giudiziario, siamo chiamati a votare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2007, n. 36, che interviene sul decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, avente ad oggetto l'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e la modifica della composizione e dei compiti dei Consigli giudiziari. Per rendere immediatamente applicabile detto decreto legislativo che recepiva la terza delle deleghe previste dalla legge n. 150, occorreva però prevedere la normativa puntuale della procedura elettorale del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e quella relativa alle modalità di svolgimento delle operazioni elettorali in rapporto delle modifiche determinate alla composizione dei Consigli giudiziari. Allo stato, però, in assenza di tale normativa puntuale, non è possibile procedere alle indizioni delle elezioni per il rinnovo dei Consigli giudiziari in scadenza il 1° aprile del corrente anno, come ci ricordava il relatore, ed è pertanto assolutamente necessario provvedere al differimento delle operazioni elettorali ed alla proroga degli attuali Consigli fino allo svolgimento delle elezioni, non essendo assolutamente ipotizzabile un'interruzione, neppure temporanea, della loro attività. Il decreto-legge del quale il Governo chiede la conversione intende, dunque, porre rimedio a tale situazione provvedendo al differimento delle elezioni e prorogando i Consigli giudiziari oggi in carica fino alla celebrazione delle nuove elezioni. Il differimento è stato circoscritto a dodici mesi, termine ritenuto sufficiente per varare la nuova normativa che disciplinerà le operazioni elettorali, come d'altra parte già previsto da un separato disegno di legge sottoposto al Parlamento: si tratta dell'Atto Senato n. 1447 del quale ho parlato prima, che all'articolo 4 disciplina, per l'appunto, questa normativa. Ecco perché il decreto-legge prevede che la scadenza dei Consigli giudiziari attualmente in carica sia prorogata fino alla proclamazione dei nuovi eletti fissando la nuova data delle elezioni per la prima domenica ed il lunedì successivo del mese di aprile dell'anno 2008. Questo è l'oggetto molto limitato del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame. Tuttavia, una considerazione, riprendendo le questioni che sono già state affrontate in Aula, ritengo che sia giusto farla. Probabilmente (e mi rivolgo al ministro Mastella), essendo già trascorso un anno dall'inizio della legislatura ed essendosi già da tempo posto il problema, il Governo avrebbe potuto essere più solerte (mi rivolgo al sottosegretario Scotti, che è molto più attento), evitando l'ennesimo intervento mediante decreto-legge. Certo, occorre ancora una volta fare di necessità virtù e prendere atto della situazione esistente. Nelle condizioni date, oggi come oggi, è evidente che non è possibile che intervenire, come sta facendo il Governo, attraverso un decreto-legge: occorreva infatti prorogare una data elettorale prevista per il 1° aprile.

cercare di intervenire prima che maturasse il termine per le elezioni e fosse necessario un ennesimo decreto-legge che in qualche modo spoglia nel momento attuale il Parlamento di una possibilità di introspezione ed è costretto nel contempo a prendere atto di una necessità che poteva essere evitata. Pertanto, non può

Se li rispetta vorrei ricordarle che nel settembre del 2006, proprio in quest'Aula e attraverso un'opera di buona volontà tra maggioranza e opposizione, così com'è stato testé ricordato anche dal collega Manzione,

relativo all'accesso in magistratura e alla professione di magistrato, non si riusciva a trovare un accordo. Con una tecnica parlamentare per me discutibile, ma che lei invece segue sempre, ha inteso rimandare l'entrata in vigore di questo decreto legislativo

Vedo che tutti cercano di distrarla, forse gli esponenti della maggioranza non vogliono che interloquiamo. sarebbe opportuno che lei venisse a seguire questo provvedimento, che è una parte importante, quasi esclusiva, dei compiti costituzionalmente previsti per il Ministro della giustizia. Non si era mai parlato di modificare questo provvedimento, un provvedimento molto importante, perché i Consigli giudiziari hanno molti compiti, che io riassumerei in uno: riassumerei in uno: sorvegliare sul buon andamento dei tribunali e degli uffici giudiziari. Noi avevamo introdotto due modifiche rilevanti rispetto all'attualità: la prima si dava più spazio all'ordine forense, in quanto gli avvocati, per unanime accordo, sono visti come uno degli elementi fondamentali dell'esercizio della giurisdizione; la seconda si prevedeva l'ingresso di esponenti del territorio, attraverso i rappresentanti delle Regioni. Ma cosa è accaduto? Nel provvedimento che adesso avete presentato al Senato, e che lei ha già dichiarato

L'ANM ha inteso, ancora una volta, statuire il suo potere sul potere legislativo. Questo è il dato fondamentale cui noi ci troviamo di fronte, nell'assoluto silenzio del Ministro, che non ho sentito ancora una volta parlare su questi temi. Parlano sempre e solo i Sottosegretari magistrati. Ma parli anche la politica! Parlino il potere legislativo ed esecutivo su questi temi! Altrimenti non si potrà far altro che prendere atto, con rammarico, che un potere

*(Ulivo)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, signori del Governo, il decreto-legge 30 marzo 2007, n. 36, del quale viene proposta la conversione in legge, concerne l'approvazione di alcune norme di proroga attinenti ai componenti dei Consigli giudiziari in carica. il 1° aprile di questo anno, cioè il giorno immediatamente successivo all'emanazione del decreto‑legge in esame, i Consigli giudiziari sono scaduti e sarebbe stato, pertanto, necessario procedere all'indizione delle elezioni per il rinnovo dei medesimi. peraltro, si sono opposte a tale indizione: da una parte, l'istituzione del nuovo Consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui al decreto legislativo 27

Allo stato, manca ancora la nuova normativa in materia. In sede di Commissione giustizia si stanno esaminando, proprio in questo periodo, le norme dell'ordinamento giudiziario che riguardano espressamente liste, composizione ed elezioni relative ai Consigli giudiziari. Ne tratta, in particolare, l'articolo 4 del disegno di legge governativo n. 1449. Non si può, pertanto, parlare in questa sede ed in questo momento di inattività del Governo, come affermato, poco fa, dal senatore Castelli.

I motivi che hanno determinato tale arco temporale sono squisitamente tecnici e sono stati adeguatamente illustrati sia nella relazione al decreto-legge che dal relatore in questa sede. L'approvazione L'approvazione del decreto-legge n. 36 si presenta, pertanto, come un atto dovuto da un punto di vista sia tecnico che giuridico, proprio al fine di evitare che, in assenza delle norme emanande, si creino situazioni di confusione o addirittura di *caos* amministrativo e funzionale in organismi indispensabili per un corretto andamento del settore giustizia a livello territoriale. In conclusione, non si può che essere favorevoli all'approvazione del testo del decreto‑legge n. 36 del 2007 che ci viene proposto.

perché tutto deve restare come prima, allora è chiaro che qualsiasi data non ha assoluto valore. Aspetto che il Ministro si pronunci su tale questione.

giustizia*. Rimbalzo nel campo del senatore Castelli: poiché il decreto-legge non è scisso e disgiunto dal disegno di legge,

Signor Presidente, intervengo a nome del Gruppo Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti italiani. II voto favorevole che il Senato si appresta a dare sull'Atto Senato n. 1449 è indispensabile per procedere al necessario differimento, in termini temporalmente contenuti, delle operazioni elettorali riguardanti i Consigli giudiziari, prorogando quelli attualmente in funzione fino alla proclamazione dei nuovi eletti. In tal modo, ovviando alle problematiche di carattere normativo e organizzativo esposte nella relazione illustrativa del disegno di legge, si consente l'adeguata organizzazione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli giudiziari presso le Corti d'appello e del Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione, organo istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, emanato in attuazione della legge delega 25 luglio 2005, n. 150. Verificata la coerenza degli aspetti tecnici normativi del decreto e delle esigenze giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari del provvedimento, dobbiamo quindi concordare con la necessità di realizzare un intervento normativo immediato, per evitare, in particolare, una temporanea cessazione delle attività dei Consigli giudiziari, che sarebbe fonte di notevole pregiudizio per il funzionamento complessivo dell'organizzazione giudiziaria e per consentire di adottare una normativa elettorale adeguata alle modifiche ordinamentali introdotte in materia. Il decreto-legge è stato, quindi, lo strumento normativo più appropriato, trattandosi di interventi necessari, urgenti e mirati, per garantire la continuità funzionale di organi collegiali elettivi aventi rilevanti attribuzioni nell'ambito dell'ordinamento giudiziario e per consentire l'introduzione nel sistema della normativa necessaria per lo svolgimento delle elezioni degli organismi interessati. Ovviamente, come è stato ribadito anche in Aula, come per ogni proroga, ci si può rammaricare del fatto che l'assenza di una normativa contenente le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali in rapporto alle modifiche apportate alla composizione dei Consigli giudiziari e all'istituzione dell'ufficio elettorale presso la Corte di cassazione ai fini della procedura elettorale abbia impedito di procedere all'indizione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli in scadenza il 1° aprile scorso. Tuttavia, va rilevato che il differimento è stato circoscritto al tempo strettamente necessario a consentire l'entrata in vigore della normativa che disciplinerà le operazioni elettorali, contenuta in un separato disegno di legge. L'impegno che il Governo e il Parlamento assumono oggi è di duplice ordine: da un lato, evitato il vuoto istituzionale, dovremo rapidamente regolamentare le mai disciplinate modalità di svolgimento delle operazioni elettorali dei Consigli giudiziari, garantendo che saranno anche svolti tutti gli adempimenti tecnici conseguenti, che riguardano soprattutto le schede da utilizzare per lo svolgimento delle elezioni. Dall'altro lato, pur trattandosi forse della parte della cosiddetta riforma Castelli su cui sono intervenute le minori osservazioni critiche, lo stesso decreto legislativo n. 25 del 2006 sui Consigli giudiziari va fatto rientrare nel novero dei temi

che deve però essere accompagnato non solo dalla rapida definizione delle regole procedimentali per le elezioni, ma anche da una riflessione più ampia sulla composizione e sul funzionamento dei Consigli,

Signor Presidente, colleghi senatori, la conversione di questo decreto legge è ulteriore passaggio, nonché tappa obbligata, del preannunciato percorso di riorganizzazione di tutto il sistema giudiziario. Non c'è da soffermarsi sui presupposti di necessità ed urgenza, circostanze lette facilmente anche dall'occhio più inesperto. Infatti, in assenza di conversione non si potrà procedere alle elezioni per il rinnovo dei Consigli giudiziari presso le corti d'appello, né del Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione. Inoltre, *nulla quaestio* sulla costituzionalità, giacché in tal senso il decreto non può suscitare alcuna valutazione, stabilendo una mera proroga senza incidere sul merito e sui princìpi di autonomia ed indipendenza delle magistrature. Il decreto altresì è titolo per garantire la costanza della funzionalità degli organi collegiali elettivi e per consentire l'introduzione della nuova procedura per le suddette Il differimento all'aprile 2008 di cui al decreto in esame - al contrario di quanto si possa obiettare - è motivo di generale intesa politica circa la congruità e la durata della proroga, anche se taluni insistono per un termine abbreviato. Del resto, non è affatto ipotizzabile una sospensione delle attività dei Consigli, che causerebbe una *vacatio* istituzionale, una violazione dei dettati costituzionali e un notevole pregiudizio alle attività giudiziarie. Dunque, il parere sul decreto-legge presentato dal ministro Mastella è senz'altro positivo, così come propizia è la strada intrapresa nell'ottica del nuovo ordinamento giudiziario. Tuttavia, se da un lato la conversione del decreto è un fatto importante, dall'altro è assolutamente fondamentale che il Governo ed il Parlamento non ritengano esaurito il proprio impegno per il ripristino e la riorganizzazione formale della struttura giudiziaria. Con questo monito, a nome dei Popolari-Udeur, esprimo voto favorevole alla conversione odierna. *(Applausi

voterà contro la conversione del decreto-legge in esame, perché sostanzialmente attendiamo di conoscere, in via definitiva, l'opinione del Governo sulla riforma dell'ordinamento giudiziario.

Ricordo soltanto che in quest'Aula abbiamo prodotto risultati utili con riferimento alle procure della Repubblica e ai procedimenti disciplinari nei confronti di magistrati. Mi auguro quindi, e il Gruppo dell'UDC lavorerà in tal senso, che si trovi un'ampia intesa istituzionale sul nuovo ordinamento giudiziario.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il voto contrario del Gruppo Forza Italia

del disegno di legge di conversione di questo decreto‑legge. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i presupposti tecnici per l'approvazione del decreto‑legge non vengono contestati. Non c'è dubbio che se il Governo resta inerte e crea una condizione di blocco, di disagio, rendendo difficile continuare ad operare, alla fine in qualche modo bisogna trovare

in senso non propriamente tecnico, ma al più basso livello - rispetto ai provvedimenti necessari per far entrare in vigore leggi che sono già leggi dello Stato. La cosa grave è il giudizio politico che bisogna dare di questa inerzia del Governo: è un'inerzia che, nella migliore delle ipotesi, prelude a cambiamenti che non possono non essere in senso peggiorativo rispetto alla riforma approvata, per quel che riguarda in particolare Siamo certi che quei piccoli passi avanti che si sono compiuti e quelle novità che sono state unanimemente apprezzate a proposito dei Consigli giudiziari, probabilmente subiranno un arretramento o saranno cancellati.

tempo necessario ad approvare le modifiche sia tempo utile a peggiorare le novità che la precedente maggioranza ha apportato in materia di giustizia. Il secondo motivo è una preoccupazione forse ancora più fondata:

l'interesse generale, un interesse generale, a mio avviso, fortemente contrario ai princìpi costituzionali. Infatti, non si può andare avanti cancellando,

contro la proposta del Governo. Signor Presidente, la proroga dei Consigli giudiziari, della quale oggi stiamo discutendo, è finalizzata al progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario che l'attuale Governo ha elaborato, che in questo momento è in discussione presso la Commissione giustizia e che dovrà essere valutato e votato dall'Aula. Io non comprendo in base a quale logica un collega, pure così avveduto e saggio come il senatore Ziccone, possa formulare un giudizio secondo cui una nuova normativa in materia di ordinamento giudiziario non può che essere peggiorativa rispetto a quella varata dal ministro Castelli e approvata in Parlamento nella scorsa legislatura. In verità, quelle norme furono il risultato di un itinerario assai complesso e contraddittorio e, se si raffrontano le norme contenute nel disegno di legge Mastella con quelle che erano proprie della prima stesura passata al Senato del testo sull'ordinamento giudiziario della scorsa legislatura, ci si accorge che i punti di convergenza sono più numerosi di quanto non siano oggi gli elementi di divergenza rispetto al testo definitivo della legge Castelli. Quella legge non solo fu respinta dal Presidente della Repubblica alle Camere, ma fu criticata da settori rilevanti della maggioranza: furono presentati emendamenti provenienti da parlamentari di Alleanza Nazionale e da parlamentari dell'UDC che, all'ultimo momento, vennero ritirati perché prevalse la disciplina di maggioranza. Allora, di fronte ad un testo di legge così criticabile e criticato, come si fa onestamente a dire: «Voi non potete che fare peggio»? E poi, voi chi? C'è una proposta avanzata dal Governo, ed è un diritto-dovere del Governo elaborare un proprio disegno di riforma di una materia che è stata così controversa.

dal Ministro della giustizia e dalle forze della maggioranza, ad avviare una discussione seria e reale per arrivare ad una nuova normativa sull'ordinamento giudiziario, come peraltro siamo riusciti a fare, sia pure in fretta stretti dal tempo, nell'autunno scorso, quando abbiamo modificato il decreto legislativo relativo all'organizzazione delle procure e quello che si riferiva al sistema disciplinare. Esistono tutte le condizioni per un dibattito serio e per la ricerca di punti di convergenza. A questo fine, la proroga dei Consigli giudiziari è un provvedimento del tutto ragionevole, altro che incostituzionalità, e che sia del tutto ragionevole è stato implicitamente riconosciuto, mi sembra, negli interventi del collega D'Onofrio e del collega Ziccone. Ci saremmo aspettati, sulla base degli argomenti di merito che pure sono stati avanzati nei loro interventi, che si manifestasse oggi una maggiore disponibilità. Comunque, noi voteremo a favore di questo provvedimento di proroga perché esso si colloca nella prospettiva di una riforma che vogliamo fare con il massimo dei consensi possibile e che riguarda il rafforzamento del circuito del governo autonomo della giurisdizione, di cui i Consigli giudiziari, articolazione territoriale di questo governo autonomo, sono un elemento fondamentale. Le valutazioni di professionalità dei magistrati, che sono così importanti per dare credibilità all'esercizio della giurisdizione, oggi non funzionano o sono insufficienti perché l'anello debole del circuito del governo autonomo della giurisdizione è rappresentato proprio dai Consigli giudiziari che sono inadeguati rispetto alla funzione che dovrebbero esercitare. La proroga serve affinché si creino le condizioni di una riforma nella quale anche i Consigli giudiziari diventino una cosa più seria, siano rafforzati e possano esperire fino in fondo le funzioni di controllo e di valutazione della professionalità che ad essi devono essere assegnate. Per tutte queste ragioni, e nella prospettiva di una riforma alla quale vogliamo lavorare seriamente nelle prossime settimane con un dibattito aperto, senza pregiudizi ma cercando di concludere presto perché i tempi stringono, voteremo a favore di questo provvedimento.

ringrazio il senatore Massimo Brutti che ha detto la verità. Lo ha testé dichiarato: la proroga serve per poter riformare l'ordinamento giudiziario. Quindi, è del tutto evidente che è vero che non c'entra nulla la questione della necessità e dell'urgenza legate al mancato varo dei regolamenti. I regolamenti non sono stati varati, appunto, per non far entrare in vigore questo provvedimento che -lo ricordo - non è mai stato criticato da nessuno:

le battaglie legate al tentativo di riforma della magistratura sono finite, non so se per stanchezza politica, se perché abbiamo perso le elezioni o se a seguito di recenti

perché non ho alcuna intenzione di immolarmi su un fronte per il quale non godo del sostegno dell'opposizione. Naturalmente, adempiremo fino in fondo al nostro dovere e voteremo contro

vorrei innanzitutto ringraziare, in questa replica alla discussione generale sul disegno di legge in materia di riordino degli enti di ricerca, tutti gli intervenuti

Emerge, oltre l'approvazione di questa legge, che spero avvenga con una maggioranza la più ampia possibile, l'esigenza di un dibattito più approfondito, evocato in molti interventi, sulla prospettiva generale del sistema di ricerca del nostro Paese, un dibattito da affrontare e che affronteremo insieme. Sono, inoltre, emersi, in molti interventi, problemi di indubbia rilevanza, ma non molto attinenti al disegno di legge in questione; faccio riferimento, in particolare, a due importanti ordini del giorno presentati dalla senatrice Pellegatta e dal senatore Davico sul precariato della ricerca.

non è una nuova legge di riordino, vorrei tranquillizzare su questo soprattutto il senatore Possa, che ha parlato di una legge di riordino fatta a due anni da una riforma generale appena conclusa.

perché il mondo della ricerca non sopporta riforme strutturali una di seguito all'altra così ravvicinate. I riordini proposti sono ben delimitati e definiti:

del giorno in Commissione anche da forze dell'opposizione; ricordo che anche nella passata legislatura sull'assorbimento dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM) ci furono molte perplessità anche all'interno di quella che è oggi la maggioranza. Quindi, noi diamo una delega al Governo, un Governo che, badate bene, dovrà raffrontarsi costantemente con le Commissioni parlamentari non per realizzare un nuovo riordino generale, ma per intervenire nei settori ben precisi, come la fisica della materia, l'ottica e l'ingegneria navale. È stata rivolta, stranamente, a questo provvedimento, anche anche una critica che io considero un po' incongrua, cioè che il Governo doveva fare una legge più articolata, più pesante, più ambiziosa. Ma, cari colleghi che avete fatto quest'obiezione, non ci sarebbe stato, in questo modo, il rischio che si facesse proprio quel nuovo riordino, quella nuova riforma generale a soli due anni di distanza che voi stessi dite di non volere?

come governare e regolare l'autonomia statutaria degli enti di ricerca, cercando di fare un passo avanti rispetto alle disposizioni contenute in questo quadro sia nella legge Berlinguer che nella legge Moratti. È indubbio che su questo era necessario fare il suddetto passo in avanti. Il mondo della ricerca che esce a seguito di queste due riforme non è affatto idilliaco e pacificato.

dire dei comitati di ricerca espressi dalla comunità scientifica che indicheranno terne di nomi, all'interno delle quali il Ministro dovrà scegliere in maniera motivata. modo non si annulla la responsabilità della politica, ma più semplicemente se ne diminuisce la discrezionalità, chiamandola a scegliere comunque su figure

Non si eliminano i comitati interni di valutazione, come nel caso del CNR, ma si coordinano i comitati interni di valutazione dei singoli enti sulla base di princìpi unitari

vale per l'Istituto italiano di tecnologia. Non viene eliminato, ma, al contrario, il senso della delega è di ricondurlo pienamente all'interno del mondo della ricerca, come del resto anche nell'ambito della discussione della passata legislatura una parte della politica, oggi all'opposizione e allora nella maggioranza, richiedeva, non per limitarne le capacità anche di internazionalizzazione, ma per farne un elemento propulsore dell'intero sistema della ricerca. Un altro problema sollevato nella discussione, al quale sono particolarmente sensibile, è relativo alla questione dei costi. Si dice che è impossibile pensare ad una riforma del sistema della ricerca ad invarianza di risorse.

l'unitarietà di intenti, pur nella diversità di opinioni che si è espressa all'interno della Commissione, l'atto in discussione potrà permettere una gestione parlamentare partecipata dello stesso esercizio della delega, pur restando essa al Governo. Il voto ampio rafforza questa prospettiva. È un elemento importante per il Senato, che dimostra una sua capacità, non solo di intervenire politicamente, ma anche di assumersi responsabilità di gestione,

di aver risposto molto prontamente all'impegno preso qui in Senato sulla base di un ordine del giorno votato da questa Aula il 23 novembre scorso, in occasione dell'approvazione della legge di conversione del decreto-legge n. 262 del 2006. Piuttosto che il regolamento di delegificazione per riordinare gli enti pubblici di ricerca, che è previsto dai commi 143, 144 e 145 dell'articolo 2 del sopracitato decreto-legge, con il provvedimento al vostro esame, che fu già presentato il 13 dicembre scorso, si ricorre invece,

approvato dal Governo. Ciò non mi esime, però, dal replicare, a nome del Governo, su alcuni punti sollevati dai senatori intervenuti durante la discussione generale. Innanzitutto, pur avendo riconosciuto poc'anzi con piacere il contributo positivo dato al testo dagli emendamenti approvati in Commissione e giudicando migliorativo anche il contributo che potrà eventualmente venire da emendamenti già presentati per l'Aula, desidero richiamare l'attenzione dei senatori sui principali punti fortemente innovativi già presenti nel testo governativo iniziale. Il primo punto è quello dell'autonomia statutaria, che mi sembra sia stato sottovalutato in alcuni interventi. La prima legge sull'autonomia delle università e degli enti di ricerca, in attuazione del dettato costituzionale, fu approvato nel lontano 1989, per iniziativa del ministro dell'epoca Antonio Ruberti.

Con questo disegno di legge, invece, sin dal primo testo, è previsto il riconoscimento agli enti dell'autonomia statutaria, ciò che il Governo giudica il principale passo riformatore e fortemente innovativo. Si tratta di un atto di fiducia nella ricerca pubblica italiana non universitaria, che riteniamo matura e capace di darsi anche le proprie autonome norme statutarie come l'università, contribuendo a coinvolgere, più e meglio, l'intera comunità della ricerca pubblica nella responsabilità strategica che essa ha per lo sviluppo del nostro Paese. Il Governo non dimentica che questo fu uno dei punti più presenti nell'ampia mobilitazione dei ricercatori contro l'ultima riforma degli enti e intende riconoscere più spazio all'esperienza diretta e specifica di ciascun ente di ricerca nella formulazione delle proprie regole, convinto che così, come si legge nel testo del provvedimento, si salvaguardi «l'indipendenza e la libera attività di ricerca, volta all'avanzamento della conoscenza», caratteristica tipica e fondante - aggiungo io - di ogni sistema pubblico di ricerca. Analoga impostazione di fondo ha avviato il Governo nel prevedere, sin dal primo testo, l'alto profilo scientifico, le competenze tecnico-organizzative dei componenti dei vari organi statutari (in particolare dei consigli d'amministrazione) e idonee procedure per la loro individuazione coinvolgenti la comunità scientifica. Vi era un'allusione implicita alle procedure ben note e diffuse nella comunità internazionale, come quella dei comitati di selezione o *search* *committee*, del resto già utilizzate dal ministro Mussi - credo - con successo nella nomina del presidente dell'Agenzia spaziale italiana. Il Governo saluta, quindi, con soddisfazione il completamento del testo originario con un'indicazione precisa ed esplicita a questa procedura, ottenuta con un emendamento approvato in Commissione. Il Governo, d'altra parte, è ben conscio che gli enti pubblici di ricerca giocano un ruolo importante nelle strategie di lungo termine del Paese e quindi saluta e giudica di nuovo con soddisfazione la possibilità, prevista in un emendamento, che il consiglio di amministrazione del

in particolare quella sulla necessità di un nuovo riordino e di un dialogo tra maggioranza e opposizione su temi come questi. Al senatore Asciutti faccio presente che questo riordino non genera costi automatici perché non tocca la struttura interna degli enti, ma solo l'autonomia statutaria e che, inoltre, prevede alleggerimenti burocratici dovuti appunto a tale autonomia. Infine, mi sembra strana, nella sua bocca, la critica al possibile scorporo dell'INFM perché, quando questo ente, ben funzionante, fu incorporato nel CNR, molti dubbi furono sollevati dalla maggioranza d'allora e anche - se non ricordo male - dal senatore Asciutti. Con la senatrice Pellegatta vorrei condividere il punto che il punto che non c'è e non ci deve essere un modello unico di *governance* degli enti e inoltre anche la necessità che si presti più attenzione alla stabilità dei rapporti di lavoro, come del resto è previsto dalla Carta europea dei ricercatori, che i senatori hanno

facilità e scioltezza e che si ponga sempre maggiore attenzione al merito e alla qualità, anche attraverso la costituenda Agenzia nazionale di valutazione che presto verrà all'esame delle Commissioni parlamentari.

sarà sempre valutata rispetto al contesto in cui si muove l'ente, com'è giusto che sia, tenendo conto anche di Regioni del Paese in cui il contesto territoriale è meno forte che in altre.

così profonde da destabilizzare gli enti. Inoltre, non mi sembra proprio che dall'attività governativa e dallo spirito meritocratico e di attenzione alla qualità con cui il Governo si è mosso in questo provvedimento, come in quello sull'Agenzia di valutazione, derivino pericoli di autoreferenzialità, anzi penso il contrario. Inoltre, senatore Possa, registro la sua contrarietà

non si tratta di spostare reparti del CNR: questo, infatti, non ha reparti, perché non è un'azienda; è un ente di ricerca che deve perseguire il bene del Paese e della conoscenza, cercando di dare a tutti il massimo spazio possibile per raggiungere i loro obiettivi.

debbo dire che, in linea di principio, il tempo per gli emendamenti è ampiamente scaduto. Ho potuto rilevare, però, una condivisione larghissima attorno a queste proposte da

del consenso me ne sono già occupato io, e c'è;

all'articolo 1, comma 4, dopo le parole: "si avvale" siano inserite le parole: ", senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato," nonché in fine siano aggiunge le seguenti parole: ", ai quali non è riconosciuto alcun compenso o indennità.";

per sottolineare, in conformità al testo costituzionale, il divieto di discriminazione di sesso, che d'altro canto è già stato affermato nella passata legislatura, ed espungere invece il riferimento al genere, che è termine sconosciuto al nostro ordinamento e persino equivoco nel dibattito costituzionale. Quindi, chiedo di mantenere un riferimento saldo alla nostra Costituzione

1.101 invito al ritiro la senatrice Pellegatta, anche perché il tema è stato in qualche modo ripuntualizzato dal subemendamento approvato

per evitare una discussione su questo tema, che non mi sembra avvenga nemmeno nella sede appropriata, è un comune richiamo all'articolo 51 della Costituzione,

l'emendamento 1.109, che mi pare di avere, se non alla lettera, colto nello spirito con l'emendamento presentato dal relatore in Aula, in cui si parla di accorpamenti e scorpori anche parziali. Non è data

1.104 vi è un invito al ritiro, perché nel caso del CNR, ad esempio, le aree di ricerca sono articolazioni territoriali e non scientifiche.

all'adozione di misure che prevedono norme antidiscriminatorie di genere nella composizione degli organi statutari. Questo dopo una bella discussione in Commissione che ha mostrato come sia l'articolo della Costituzione sia altre diciture siano più arretrate rispetto al dibattito del movimento delle donne in Europa e in Italia, in cui non si usano più tali termini e non a caso, in quanto si considera il genere

Signor Presidente, colleghi senatori, promuovere la ridefinizione degli enti di ricerca è cosa impellente. Infatti, l'intento di riordino avviato dai precedenti Governi non è stato sostenuto adeguatamente da atti di indirizzo, sicché la vita degli stessi è stata condizionata da logiche politiche. Ora, viceversa, è tempo di superare le scelte strumentali precedenti e riconoscere il primato al principio di autonomia scientifica. Adesso l'impegno del Governo è per una ricognizione totale degli enti vigilati dal MIUR (Ministero dell'università e della ricerca): una ristrutturazione che può prevedere anche l'accorpamento, la fusione e la soppressione degli enti stessi, ma che comunque dovrà incrementare le capacità di monitoraggio e valutazione della ricerca. Promuovere l'autonomia di questi enti significa, soprattutto, sviluppo di attività comuni finalizzate all'impegno produttivo delle conoscenze e incentivo alle interazioni con le università. Tale nuovo *input* assicurerà spazi adeguati all'irrinunciabile attività di ricerca, intesa anche al servizio del mondo produttivo, cosicché si realizzi una sistematica cooperazione con le imprese e si abbandoni l'antico retaggio di relazioni opportunistiche. Nel nuovo apparato si esalterà il ruolo della ricerca per gettare le basi di un sistema «Qualità Italia» che incrementi la competitività del Paese e costituisca un polo organizzato nei nuovi segmenti di mercato: dunque più autonomia e più caratterizzazione dei rispettivi compiti al fine di incrementare il monitoraggio e lo sviluppo della ricerca. Per questi motivi, a nome del Gruppo dei Popolari Udeur, esprimo voto favorevole al disegno di legge in esame.

Fare presto e fare bene: era questo l'auspicio che abbiamo espresso quando abbiamo avviato il confronto su questo provvedimento in materia di riordino degli enti di ricerca in 7a Commissione. Fare presto era una necessità per diversi motivi: da un lato, il cattivo stato di salute di alcuni enti; dall'altro, l'evidenziarsi di urgenze di fronte ad importanti occasioni che l'Europa mette a disposizione della ricerca. Sarebbe assolutamente colpevole non cogliere le opportunità previste dal VII Programma quadro dell'Unione Europea. Dopo pochi mesi, con nel mezzo momenti difficili per la vita parlamentare, come la crisi di Governo, arriviamo a licenziare il testo. Credo che possiamo dirci soddisfatti: abbiamo usato il tempo necessario, senza sprechi, per una materia molto complessa e crediamo anche, rispetto alla necessità di fare bene, che il testo che consegniamo alla Camera sia migliore e più puntuale della già ottima base di discussione che il Governo ha consegnato al Senato. La discussione approfondita che abbiamo affrontato, tanto in Commissione come in quest'Aula, porta a migliorare il testo. Ma, a fronte di alcune critiche ingenerose ascoltate in discussione generale, credo sia utile dare atto della sensibilità dimostrata dal Governo, che ha scelto la corretta via della delega legislativa sospendendo l'uso della delega regolamentare prevista in finanziaria e spronando il Parlamento a farsi carico di una scelta più puntuale e complessiva. Oggi, grazie a questo provvedimento, la scienza del nostro Paese sarà più libera e autonoma. Crediamo sia utile, allora, mettere in luce alcuni elementi che, grazie all'impegno di tutte le forze politiche, rafforzeranno l'autonomia e la produttività degli enti di ricerca. L'introduzione dei *search committee* consente di affermare con forza che la competenza scientifica e gestionale sono criteri sovraordinanti alle appartenenze e alle sensibilità: è un primo passo, importante, per rafforzare davvero il nostro sistema della ricerca, superando inaccettabili nepotismi. Un secondo aspetto che ci sembra utile salutare con soddisfazione è la puntualizzazione nell'identificare quegli enti e quelle strutture che necessitano dei maggiori interventi: il rilancio della ricerca nei settori dell'ottica e della fisica della materia sono obiettivi che spero possano essere da tutti condivisi. Così come il riferimento alla Carta europea dei ricercatori ci sembra una scelta utile, se non sarà un semplice orpello. Ma vogliamo ricordare a tutti cosa prevede questa Carta citiamo solo tre princìpi che lì sono contenuti: gli enti devono offrire condizioni di lavoro che consentano sia alle donne sia agli uomini di conciliare famiglia e lavoro, figli e carriera; gli enti devono riconoscere la necessità che i ricercatori siano rappresentati negli organi decisionali; gli enti devono garantire che le prestazioni dei ricercatori non risentano dell'instabilità, ma anzi devono operare per migliorare la stabilità delle condizioni di lavoro dei ricercatori. Sono tre passaggi estremamente impegnativi che disegnano un mondo della ricerca dove il ruolo dei ricercatori sia anche quello di decidere del futuro del proprio lavoro, in un contesto di piena autonomia scientifica, garantito dalla stabilità del rapporto di lavoro. E proprio la Carta europea ci sollecita, rispetto all'enorme questione di genere che investe gli enti di ricerca, a non limitarci a sole misure prescrittive, ma a costruire politiche attive per le pari opportunità; è questo, allora, che ci aspettiamo dal Governo in quest'opera di riordino: la capacità di garantire la conciliabilità dei tempi di vita e di lavoro come un elemento necessario per liberare le energie delle nostre ricercatrici e ricercatori. Ma questi interventi richiedono ed esigono di affrontare con decisione altre due questioni che completino il quadro: l'estensione di questo approccio al complesso della ricerca e l'impegno economico del Paese verso la ricerca. Se, nella classifica mondiale delle imprese più innovative, la prima azienda italiana, abbastanza isolata, è Finmeccanica, al cinquantesimo posto, questo è sicuramente dovuto alla parcellizzazione del nostro sistema produttivo e ai limiti del nostro capitalismo, ma è in parte dovuto anche alla debolezza del nostro sistema di ricerca, debolezza non solo e non tanto nella produzione scientifica, ma anche nella capacità di trasmettere i risultati di questo impegno alla ricerca applicata, e alla debolezza del sistema delle imprese di assumere quei risultati come *asset* strategici. Se questi sono i dati, serve fin dalla prossima legge finanziaria un impegno straordinario: la scelta da parte del Governo di porre la ricerca tra le assolute priorità, confermata nel corso del recente riconsolidamento della maggioranza con il cosiddetto dodecalogo, deve avere effetti anche sul bilancio dello Stato. L'altro punto aperto all'iniziativa del Governo e del Parlamento, come già registrato dal relatore nella discussione generale, resta quello degli enti di ricerca che non dipendono dal Ministero dell'università e della ricerca: vi sono decine di luoghi pubblici dove la ricerca potrebbe essere un elemento trainante dello sviluppo, ma che sono lasciate senza forma forma alcuna di coordinamento e dove anche le condizioni di lavoro dei ricercatori sono estremamente diseguali. Solo per citare tre esempi di prima grandezza, pensiamo all'ISTAT, che sta affrontando una complessa transizione da ente pubblico a ente di ricerca, o ancora all'ENEA, dove vige un curioso contratto che non esiste in nessun'altra struttura italiana e che deve anch'esso chiarire la propria missione strategica, o a situazioni assurde e incomprensibili, come quella del Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura, il CRA, dove i ricercatori hanno il contratto da braccianti. È necessario e urgente, allora, che il Governo tutto superi l'atteggiamento dei compartimenti stagni, per cui i singoli enti di ricerca sono riserva di ciascun Ministero. Siamo convinti che, a partire dalla valutazione, forme di coordinamento, procedure standardizzate e rapporti di lavoro omogenei, pur nel rispetto dell'autonomia della scienza, darebbero un forte impulso al nostro sistema scientifico, così come siamo fiduciosi che il clima che ha accompagnato il nostro lavoro in Commissione possa confermarsi. Pur rimanendo una perplessità sulla scelta di preordinare il ruolo dei consigli di amministrazione, per tutto quanto detto sopra dichiaro il voto favorevole del Gruppo Insieme con l'Unione

Signor Presidente, colleghi e colleghe, la legge delega che ci accingiamo oggi ad approvare è un primo concreto passaggio di un percorso che ci dovrà portare a una politica della ricerca adeguata alle esigenze di questa fase storica e, soprattutto, al bisogno impellente, per il nostro Paese, di superare un vero e proprio stato di minorità, in Europa e nel mondo. Noi di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea la voteremo con questa convinzione e con questa consapevolezza, sapendo, cioè, che si tratta solo di un primo passo per superare le inerzie, le resistenze e le opposizioni che, al di là delle dichiarazioni di intenti o degli impegni verbali, non ci consentono ancora di puntare sulla ricerca - e sulla ricerca di base - come volano privilegiato per uscire dal rischio di declino che ci minaccia; sapendo che ancora pesa, ben al di là della volontà di chi governa e dei Ministri competenti, un'idea, diciamo così, contabile e quantitativa della crescita, del lavoro produttivo, dell'impiego delle risorse. Prendiamo atto, dunque, che con questa proposta si mettono alcuni degli enti della ricerca pubblica più importanti, quelli direttamente vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, in condizioni nettamente migliori che nel loro, peraltro accidentato, passato. legislativa finale, che è stata notoriamente il frutto di un vero e lungo dibattito in 7ª Commissione, apprezziamo, in particolare, l'equilibro raggiunto tra la necessità dell'autonomia degli enti e la necessità analoga di un rapporto positivo e non condizionante con la politica. In realtà, dentro questo problema - così come ha rilevato in sede di discussione generale la nostra collega Capelli - si cela una questione di straordinaria complessità culturale: cos'è la libertà della ricerca nell'epoca della globalizzazione e di uno sviluppo della scienza senza precedenti? Chi decide, con quali criteri, con quali paradigmi, con quali possibilità di valutazione, con quali risultati? Non credo che nessuno possa cavarsela, su questi temi, con ricette semplici. Credo però che, intanto, possiamo approssimarci a questi a questi problemi tenendo ferme due barre: per un verso, è essenziale l'autonomia dei soggetti che la ricerca la compiono ogni giorno sul campo; per altro verso, è quasi altrettanto essenziale che la politica - intesa nel senso più lato e alto del termine - svolga un ruolo di indirizzo, garanzia, stimolo, controllo critico. La politica che non può esaurirsi nella dimensione del Governo e che perciò, come sta scritto in questa legge, comprende attivamente il lavoro del Parlamento e dovrà, secondo noi, riuscire a coinvolgere altre istanze democratiche e rappresentative della società. Fino a qui vale il nostro consenso, quello che ci spingerà a votare a favore di questa legge. Adesso vorrei solo dedicare l'ultima parte della mia dichiarazione di voto ad un punto serio di dissenso che abbiamo dovuto registrare durante la discussione e la votazione degli emendamenti. Il fatto che la dizione sulle norme antidiscriminatorie di genere sia stata modificata con il ritorno alla dizione originaria del testo di legge, che avevamo modificato dopo un un interessante ed approfondito dibattito in seno alla nostra Commissione, ci lascia l'amaro in bocca. Vorrei spiegare ai colleghi che hanno preferito tornare a quella dizione che non solo il linguaggio non è neutro, ma che la discriminazione di sesso e la discriminazione di genere e la stessa dizione delle pari opportunità non significano affatto la stessa cosa: in ogni caso, la dizione «norme antidiscriminatorie di genere» non si riferisce più ad una differenza di tipo biologico-naturalistico e che in qualche modo ci riconduce a quella pretesa incompatibilità tra donne e scienza che è corsa per tanto tempo nella nostra cultura; la discriminazione di genere ha un senso diverso e richiama anche un tema difficile e duro com'è quello non solo del rapporto

collocazione, anche da questo punto di vista, nei riguardi del genere maschile e della sua tendenza a perpetuare il patriarcato. Ricordo qui che addirittura stiamo parlando di una situazione di cui non si può non prendere atto: in una struttura significativa come l'ENEA, un'inchiesta svoltasi l'anno scorso dimostra che le donne sono discriminate sul piano non solo delle carriere, ma del salario e guadagnano mediamente il 30 per cento in meno dei loro colleghi maschi, naturalmente a parità di qualifica.

voteremo, con disappunto, l'insieme di questa legge che ci sta a cuore, ma ci impegniamo e contiamo sul fatto che sulla specifica questione delle norme antidiscriminatorie la Camera possa correggere quello che noi qui al Senato non siamo non siamo riusciti a fare, nella speranza di poter tornare a discutere, con reciproco rispetto, profitto e comprensione, di un tema di questa portata.

aveva tentato già in passato una ridefinizione della missione e il conseguente riposizionamento degli enti di ricerca. Tale riordino non era stato supportato da adeguati atti di indirizzo, sicché l'autonomia degli enti si era espressa su scelte di carattere politico-strategico che hanno, in taluni casi, leso il principio dell'autonomia scientifica. Ciascun ente, di conseguenza, si è trovato immesso in logiche autoreferenziali e teso a conservare l'insieme di funzioni ed attività ereditate dal passato. Anche in quest'occasione, il Governo di centro-sinistra ha rischiato nelle settimane scorse di fallire, procedendo al riordino degli enti attraverso regolamenti di delegificazione che avrebbero minato la tutela legislativa dell'autonomia degli enti di ricerca, che trova il suo fondamento nell'articolo 33 della Costituzione, e creato contenziosi tra lo Stato e le Regioni, dal momento che l'articolo 117 della Costituzione affida alla competenza concorrente la materia relativa alla ricerca. L'operazione, che inizialmente questo Governo ha cercato di attuare, non sembrava sorretta da una strategia efficace, volta al rilancio della ricerca pubblica italiana, il cui obiettivo deve tendere alla valorizzazione del personale scientifico che in essa opera. Pur esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto in Commissione, grazie alla presidente, senatrice Franco, e alla disponibilità del relatore, senatore Ranieri, che ha contribuito a stabilire i giusti princìpi e criteri direttivi, non configurati nel testo originario del disegno di legge, tanto da far sospettare, come già ribadito in sede di discussione generale, che il Governo volesse commissariare la ricerca italiana, rimangono alcune perplessità sul tenore di un provvedimento che non chiarisce alcuni aspetti. Infatti, se da un lato va registrata positivamente l'introduzione di un esplicito richiamo alla Carta europea dei ricercatori; del riconoscimento, in linea di principio, di un'autonomia anche statutaria degli enti; della previsione che i direttori delle strutture scientifiche debbano essere scelti tramite procedure di valutazione comparativa sulla base del merito scientifico della nomina dei comitati di selezione di rose di candidati alle presidenze, dall'altro, mancano raccordi con l'autonomia regionale (nel testo si fa riferimento ad eventuali attività d'interesse delle Regioni) la scarsa attenzione al mondo imprenditoriale nonché la vaghezza su eventuali nuovi incentivi o risparmi derivanti dal nuovo assetto degli enti. Si invoca la libertà di ricerca, pur essendo consapevoli che detta attività dipende, in misura preponderante, da finanziamenti esterni, in larga misura privati, che condizionano necessariamente l'indipendenza nello svolgimento dell'attività di ricerca. A questo proposito giova ricordare che le dotazioni ordinarie stanziate dalla finanziaria 2007 si sono ridotte a livello di pura sussistenza, laddove dovrebbero essere assicurate per il buon funzionamento delle strutture di ricerca e lo sviluppo di conoscenze e competenze non immediatamente applicabili. Il caso INAF è davvero emblematico. Il taglio del 5 per cento dei fondi ha significato di fatto tagliare un quinto della ricerca. Il 75 per cento dei fondi è impiegato per il pagamento del personale, sovradimensionato rispetto a chi svolge attività di ricerca. Milioni di euro sul bilancio dell'ente per gli incomprimibili stipendi di 50 impiegati amministrativi, di cui non hanno mai usufruito osservatori e centri esterni all'ente stesso. Una situazione disastrosa, causata da un problema di incomunicabilità tra consiglio d'amministrazione e consiglio scientifico. La conseguenza è la chiusura del telescopio nazionale «Galileo» alle Canarie, l'impossibilità di pagare addirittura l'ultima rata del progetto internazionale «*Large binocular telescope*», al quale l'INAF partecipa da dieci anni e che diventerà, a breve, operativo in Arizona, l'abbandono del radiotelescopio in Sardegna, il blocco di decine di ricerche e progetti già iniziati. La vicenda INAF è solo l'ultima in ordine di tempo. Basti pensare all'ASI, all'IMONT (l'Istituto per la montagna), recentemente commissariato e, infine, al CNR, il cui sistema fortemente burocratizzato ha creato una catena gerarchica sorprendente. Per quanto attiene ai criteri di valutazione in termini di produttività ed efficienza, bisogna tener conto che i parametri di quantizzazione, adatti a classificare i soggetti di ricerca con un giudizio di merito, espresso da uno o più indici numerici, sono validi solo se riferiti al lungo periodo. L'analisi di capacità di ciascun ente di rispondere alla missione assegnata è strettamente connessa con gli strumenti propri dell'autonomia organizzativa e scientifica. La valutazione del grado di conseguimento degli specifici obiettivi e del loro «ritorno», ad effettivo beneficio delle esigenze sociali che attraverso essi si intenda soddisfare, può avvenire «*a posteriori*», non prima di otto-dieci anni. Le parole d'ordine per il successo della ricerca si identificano con i princìpi di «produttività, massa critica e capacità di autofinanziamento». La produttività di un ricercatore o di un gruppo di ricercatori è un concetto strettamente associato a quello di efficienza. Questi criteri implicano una maggiore attenzione sui grossi gruppi, particolarmente utili, specie se fanno un lavoro in rapporto adeguato ai mezzi che hanno a disposizione ed avendo per finalità principale gli interessi della scienza e del Paese. I grandi gruppi importanti sono utili, ma riteniamo che non bisogna differenziare per ruolo, né per temi programmatici, i gruppi di minore dimensione. La dura realtà è che il Paese Italia è costituito da laboratori e piccoli centri di ricerca dotati di una strumentazione praticamente obsoleta e situati in aree di ricerca che costano più di quanto si possa spendere. Gli scienziati sono di età media e costretti a confrontarsi con finanziatori privati che, specie quando si tratta di imprese, troppe volte non hanno la giusta sintonia e la giusta considerazione della ricerca pubblica. Né vi sono posti di lavoro a tempo indeterminato paragonabili a quelli di cui dispongono gli scienziati di altri Paesi. Una legge delega che interviene, operando per la terza volta in dieci anni lo scorporo e la fusione di enti di ricerca, rischia di determinare come osservato dalla Corte dei conti e da illustri gerarchie degli enti medesimi - dispersione, piuttosto che consolidamento dell'attività scientifica. L'ultima relazione della Corte dei conti spiega che al CNR il 94,9 per cento dei fondi del Ministero sono stati impiegati per il pagamento degli stipendi. Il personale è diminuito del 10 per cento (758 unità in meno), eppure i costi sono cresciuti del 5 per cento (22 milioni di euro in più). Questo paradosso è determinato dalla politica della buonuscita e dagli scatti automatici: ogni persona che va in quiescenza costa, per quell'anno, all'ente, come tre persone di pari livello del quiescente. Il contributo alla ricerca propositiva, secondo la Corte dei conti, è diminuito del 25 E, qualora fossero vere le notizie apparse recentemente sui *media*, risulterebbe tragicomica la posizione di importanti e qualificati dirigenti. Gli obiettivi principali del riordino degli enti di ricerca si identificano con il rilancio della ricerca attraverso determinate azioni. In ogni caso, non dobbiamo comunque dimenticare che il principale prodotto dell'attività di ricerca non va individuato solo nella solo scoperta in sé, ma anche nella figura del ricercatore, indispensabile per il conseguimento dell'innovazione scientifica, poiché per creare la ricerca è necessario un lungo processo di apprendimento. In ogni caso l'attività di ricerca è importante, in quanto consente di elevare la qualità della struttura sociale che costituisce la cornice, diffondendo la percezione dei fondamenti scientifici e tecnologici delle società moderne. In sintesi, la conclusione è che questa legge delega non riesce ad andare al di là dell'ingegneria istituzionale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione generale e l'esame degli emendamenti hanno confermato la previsione che già esprimevo in sede di discussione generale qualche settimana fa. L'accordo sul testo, così come era stato liquidato dalla 7a Commissione, viene confermato dall'Aula. Abbiamo lavorato in modo intenso, puntuale ed efficace. L'UDC rivendica per sé un ruolo attivo e propositivo nella stesura condivisa del testo definitivo. La prima dimostrazione di ciò è data dal bassissimo numero di emendamenti. Riguardo a questi, ne restava uno che doveva chiarire un aspetto importante, relativo all'introduzione di una norma antidiscriminatoria di genere nella selezione degli amministratori degli enti di ricerca. Ritenevamo infatti inutile l'inserimento di questa specificazione, visto che la stessa Costituzione della Repubblica e infinite altre leggi escludono in modo perentorio qualsiasi forma di discriminazione che faccia riferimento alla razza, al sesso o a qualsiasi altro criterio di natura politica, culturale e territoriale. Quindi, il principio è saldamente stabilito ed ancorato nel nostro sistema legislativo. Pertanto, l'emendamento presentato dalle colleghe di Rifondazione Comunista ci era sembrato superfluo, comunque inutile ai fini pratici. Nonostante ciò abbiamo accolto l'ipotesi di inserire questo principio dell'antidiscriminazione facendo, però, esplicito riferimento al sesso e non al più equivoco termine di «genere», del quale riteniamo si stia facendo un certo abuso. Nel merito del provvedimento non ho altro da puntualizzare. Il nostro voto favorevole è esclusivamente legato al giudizio su questo specifico testo di legge e sul modo in cui siamo arrivati a definirlo. Il testo ci soddisfa sul piano del contenuto. Abbiamo una legge equilibrata, che fissa chiari princìpi riguardo al sistema di regole che devono disciplinare l'autonomia degli enti di ricerca, tenendo dentro confini ben delineati l'intervento della politica. Questa agisce attraverso le istituzioni (Parlamento e Governo), esercitando l'insostituibile attività di programmazione e di controllo. Il controllo diventa soprattutto, con questa legge, una verifica dei risultati. Se é importante, infatti, un attento esame dei progetti, è ancora più importante e decisivo verificare il prodotto finale. Questo non è lesivo dell'autonomia. Tutta l'autonomia ai ricercatori nel definire modalità, procedure, metodi e tempi dei loro progetti; questo è fuori discussione e su questo terreno non potranno essere tollerate ingerenze. L'UDC teneva in modo particolare che sia gli obiettivi che i risultati fossero stabiliti dal Governo e dallo stesso puntualmente verificati. Qui vediamo salvaguardato il primato dell'interesse pubblico su qualsiasi spinta corporativa o lobbistica. Il filtro e il discernimento riguardo a questi dev'essere fatto dalla politica, in questo caso dal Governo controllato dal Parlamento. Altro aspetto riguarda la modalità di composizione dei consigli d'amministrazione. Le norme previste danno un senso più chiaro al confine fra gestione e indirizzo politico. L'aver accettato questo principio da parte della maggioranza e del Governo crediamo sia stato un altro segnale importante del dialogo che ha portato a un testo largamente condiviso. È importante che, per il momento, ci diamo criteri condivisi nel fissare le regole con le quali si applicherà l'autonomia di gestione. In un secondo tempo sarà importante riscontrare la sincerità del Governo riguardo alle nomine che verranno fatte. Non possiamo, infatti, dimenticare quanto il ministro Mussi ha in proposito dichiarato in Commissione: nessuna volontà di usare lo strumento del riordino per tagliare teste ai vertici degli enti di ricerca. Una dichiarazione importante, questa del Ministro, che ci ha rassicurato per le future designazioni e, alla quale diamo credibilità. Queste nomine dovranno essere fatte secondo criteri di pura professionalità, come previsto dal punto *f*), comma 1, dell'articolo punto *f*), comma 1, dell'articolo 1, che abbiamo dovuto introdurre. L'UDC ha criticato pesantemente il modo in cui anche questo Governo ha adottato il sistema delle spoliazioni. Attraverso questo si buttano a mare alte e preziose professionalità maturate faticosamente nel tempo, solo perché la nomina è stata fatta da un precedente Esecutivo. Crediamo che il buon senso debba ritrovare una sua collocazione adeguata nell'azione politica dei partiti e degli schieramenti. Vogliamo avere fiducia che le cose possano cambiare in questa direzione e la pubblica amministrazione trovi una sua oggettiva stabilità per l'evidente vantaggio di ogni cittadino. L'amministrazione degli enti di ricerca, più di altri settori della pubblica amministrazione, per gli alti obbiettivi a cui è deputata, non può essere un terreno di scontro fra partiti o gruppi di interesse. Altro passaggio decisivo nel merito della legge riguarda l'obbligo per gli statuti degli enti di essere sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti e il fatto che il Governo potrà procedere al commissariamento degli enti attraverso decreti sempre e comunque sottoposti al parere delle Commissioni. Vediamo in questi passaggi evidenti limiti alla stessa legge delega. L'ultima questione riguarda proprio l'appoggio che stiamo assicurando a una legge delega del Governo. In Commissione avevamo chiesto di arrivare a un nuovo disegno di legge presentato da tutti i Gruppi, visto che i contenuti erano stati largamente condivisi e la legge entra in modo ampio su tante questioni precedentemente non previste dal testo del Governo. Queste iniziali carenze forse giustificavano la stessa legge delega, ma l'averle definite in Commissione dava dava la possibilità di far cadere questa necessità prioritaria. Non è stato possibile farlo; il Governo ha voluto mantenere il proprio disegno di legge delega, ma su questa strada comunque ci eravamo incamminati e tutti i Gruppi, di maggioranza e di opposizione, hanno lavorato di comune accordo per proporre un consistente pacchetto di emendamenti, concordati col relatore e col Governo, che hanno prodotto una legge sostanzialmente diversa dal testo originario presentato dalla maggioranza. Questa non è appena una nostra opinione, ma è l'evidenza che ogni collega senatore può facilmente verificare: basta confrontare il testo proposto dal Governo e quello che l'Aula si appresta a votare questa sera. Tutto ciò è per noi sufficiente per esprimere un voto favorevole, come abbiamo già fatto in Commissione. Non possiamo, d'altra parte, dimenticare che, all'inizio dell'*iter* del provvedimento di legge in esame, si era parlato con insistenza dell'intenzione dell'Esecutivo di procedere a colpi di decreto ministeriale per il riordino degli enti di ricerca. Rispetto a quella sciagurata partenza, credo che l'UDC abbia svolto un ottimo lavoro, che ha portato - lo ribadisco ancora una volta - alla quasi totale condivisione della legge nel merito dei suoi contenuti da parte di tutti i Gruppi del Senato. Da ultimo, il nostro convincimento positivo viene confermato per una volontà comune - espressa dall'ordine del giorno precedentemente votato - che sta emergendo a favore del finanziamento della ricerca,

per impegnare il Governo a presentare leggi finanziarie che prevedano un progressivo e significativo aumento dei capitoli di bilancio riservati alla ricerca. L'UDC vigilerà attentamente nel futuro perché questo orientamento sia confermato sotto ogni aspetto formale e, soprattutto, che la consistenza di questo innalzamento degli stanziamenti sia sufficiente per far raggiungere, prima della fine della legislatura, un livello di finanziamenti alla ricerca pari a quello degli altri Paesi dell'Unione Europea. In conclusione, su questo tema così caro e strategico per l'interesse del Paese, siamo orgogliosi di aver fornito un contributo decisivo e positivo, che, una volta tanto, è stato capace di mettere da parte l'interesse di bottega per dare al Paese una buona legge capace di rilanciare la ricerca.*(Applausi

che, con buona pace della sinistra radicale, i decreti Moratti non sono stati abrogati e sono stati, anzi, richiamati come legge vigente proprio nella parte sul commissariamento. Nel disegno di legge si afferma poi con chiarezza il carattere strumentale degli enti di ricerca rispetto alle politiche di sviluppo strategico delineate dal Governo. Il potere di Governo degli enti è rimasto saldamente nelle mani dei consigli di amministrazione e non dei Consigli scientifici: chiamatela logica aziendalista; noi la chiamiamo logica e basta. Desidero anche sottolineare che in nessun passaggio del disegno di legge si prevede l'eliminazione dei membri esterni, quelli che esprimono le istanze del mondo produttivo; anzi, implicitamente si stabilisce che una parte dei comitati di selezione per la composizione dei consigli di amministrazione sarà espressione della società civile, là dove si afferma che occorre assicurare negli stessi comitati un'adeguata rappresentanza di esponenti della comunità scientifica. vuol dire, dunque, che questi sono una parte, non la totalità. D'altro canto, voglio ricordare che nel consiglio di amministrazione del CNRS francese sono scelti dal Governo esponenti del mondo economico e produttivo: questo, in Francia, viene considerato un arricchimento. Di diverso tenore l'intervento della senatrice Negri, che devo tuttavia correggere su un punto non secondario: non è vero che il disegno di legge governativo contenesse già *in* *nuce* quanto poi l'opposizione avrebbe esplicitato; non vi era nulla sulla valutazione, così come non vi era nulla sugli obiettivi fissati dal Governo, né sul commissariamento nel caso di un loro mancato raggiungimento;

elettive dei presidenti degli enti e dei direttori di istituto; qui si valorizza il ruolo della comunità scientifica, ma escludendo che presidenti o dirigenti possano essere eletti: è l'ipotesi anglosassone del *search* *committee*. Più articolata deve essere, invece, la risposta all'intervento dell'amico Possa, di cui ho molto apprezzato alcuni passaggi. Premetto, come ho già sottolineato, che i decreti Moratti non vengono abrogati ed essendo legge vigente non potranno essere derogati dagli statuti. Dunque, era già implicita nel testo arrivato in Aula una netta separazione fra consiglio di amministrazione e consiglio scientifico: l'attribuzione al consiglio scientifico di compiti di governo, essendo estranea al sistema, avrebbe dovuto essere prevista tra i criteri direttivi per poter caratterizzare i decreti e gli statuti. Oggi, su nostra richiesta, abbiamo votato un emendamento - accolto dal relatore il quale si è introdotta un'ulteriore precisazione che rende esplicita la distinzione tra consiglio di amministrazione e comitati scientifici, ribadendo espressamente la continuità con i decreti Moratti. Al di là di ciò, io credo che questa legge contenga due princìpi importanti, senz'altro nuovi, e un terzo principio che è obbligato. Innanzitutto, i nuovi criteri di nomina dei presidenti e di parte dei consigli

L'autonomia statutaria - terzo principio importante - è prevista nella Costituzione e ad essa noi ci siamo più volte richiamati, per esempio, proprio per affermare la incostituzionalità dei commi 143 e seguenti del famigerato decreto fiscale qui abrogati. Trovo, dunque, positiva l'autonomia purché sia delimitata da robuste garanzie e anche a questo proposito sono stati introdotti nel passaggio parlamentare per merito dell'opposizione paletti ben fermi: intanto i presidenti degli enti sono tutti di nomina governativa, pur con le nuove procedure di selezione (per il CNR la situazione non varia rispetto alla situazione attuale), e le modifiche statutarie devono poi essere approvate dal Ministro, sentito il parere obbligatorio del Parlamento. Non solo. Credo sia sacrosanto anche un altro elemento introdotto con un ulteriore emendamento dell'opposizione e del tutto estraneo al progetto di Mussi: gli obiettivi specifici di ogni ente li fissa il Governo e se non vengono raggiunti raggiunti il consiglio di amministrazione può saltare. Ciò riecheggia la legge francese che definisce il CNRS un organismo di ricerca finanziato dal Governo e, dunque, sottoposto all'autorità amministrativa del ministro della ricerca francese. Non a caso anche in questo disegno di legge, come già nei decreti Moratti, si parla di «enti vigilati». Del resto gli enti pubblici di ricerca, a differenza delle università che hanno un'altra tradizione, si giustificano in quanto - come è scritto nelle leggi istitutive - hanno lo scopo di promuovere e coordinare la ricerca al fine del progresso della scienza e della tecnica; hanno, quindi, lo scopo di potenziare l'azione generale di governo. Nelle leggi coeve alla Costituzione repubblicana che provvidero alla rifondazione del CNR si parlava espressamente di organi dello Stato. È giusto, pertanto, che i soldi pubblici non vengano spesi per compiacere curiosità personali: se le ricerche sulla riproduzione delle farfalle non verranno giudicate fra gli obiettivi strategici dal Governo, non verranno finanziate. In questo quadro è corretto, invece, che il Governo si assuma la responsabilità di indicare specifici obiettivi come, per esempio, lo sviluppo delle ricerche nel campo delle nanotecnologie o lo studio dei legami culturali fra le due sponde del Mediterraneo. All'interno di questi elementi di controllo, l'autonomia statutaria è un contributo positivo: può garantire una maggiore flessibilità, una maggiore adeguatezza dell'ente per il raggiungimento degli obiettivi. Un contributo di esperienza che venga dall'interno dell'ente su come meglio svolgere le proprie funzioni e nei limiti indicati, ritengo sia senz'altro utile. Grazie agli emendamenti dell'opposizione, l'autonomia non è affatto autoreferenzialità. Avrebbe corso il rischio di esserlo senza i nostri emendamenti, con vertici irresponsabili e la possibilità di presidenti eletti dalla base. Autonomia e responsabilità sono ora i due princìpi cardine di questo disegno di legge. Nel testo del Governo c'era solo l'autonomia senza la responsabilità. Nel dibattito in Commissione sono stati poi respinti tutti gli emendamenti di una parte della maggioranza che, per esempio, puntavano alla elettività degli organi direttivi, al ruolo gestionale dei consigli scientifici, all'assunzione di personale non tramite concorso. Persino sul tentativo di introdurre nel nostro ordinamento il concetto di genere, anziché di sesso, in materia di divieto di discriminazioni l'opposizione ha fatto sentire efficacemente la sua voce. Certo, noi e Mussi abbiamo idee diverse (lo si è visto in tutto il percorso), ma per come abbiamo giocato il nostro ruolo in Commissione ne è uscito un testo i cui princìpi sono condivisibili. Dunque, abbiamo fatto bene a dialogare. Avendo noi a cuore l'interesse nazionale, non avevamo altra scelta. Potevamo ritirarci sull'Aventino e lasciare che una composita maggioranza introducesse princìpi pericolosi per la ricerca italiana per poi passare a riscuotere, in termini propagandistici, inveendo contro la inadeguatezza di questo Governo, oppure potevamo cercare di condizionare il testo. Abbiamo scelto questa seconda strada e il risultato è stato ampiamente positivo. Ne siamo legittimamente soddisfatti perché, cari colleghi, da questa legge non si gioca il destino del Governo Prodi, ma da una cattiva legge poteva giocarsi una minore competitività del Paese e, dunque, il suo destino. Ora che fare? Se non ci trovassimo di fronte ad una legge delega non avremmo avuto dubbi: questo testo l'abbiamo riscritto noi come opposizione. Tuttavia, si tratta di una delega ad un Governo che in questi mesi ha evidenziato differenze culturali e programmatiche troppo forti perché si possa dargli mandato di attuare con norme di dettaglio i princìpi che qui noi abbiamo fissato. Soprattutto non ci è piaciuto l'atteggiamento su un altro settore strategico, quello dell'università. Proprio pochi giorni fa la Corte dei conti ha bocciato il decreto Mussi sugli ordinamenti didattici universitari: si è trattato di una bocciatura dettagliata, articolata, profonda che ha dimostrato come ci si trovi di fronte ad un Governo pasticcione che riesce a combinare guai anche sulle norme di dettaglio. Non ci è nemmeno piaciuto che sull'ANVUR non si sia aperto nessun confronto con la opposizione e che la pessima riforma relativa al reclutamento dei ricercatori non passerà attraverso un dibattito parlamentare aperto e approfondito, ma si farà tutta a livello di decreti governativi. Caro Ministro, noi intendiamo proseguire il dialogo iniziato con questo disegno di legge anche per quanto riguarda la stesura degli statuti degli enti: decideremo alla fine se votarli o no. Per ora, pur apprezzando il testo per come è emerso dopo una profonda attività emendatrice, non ce la sentiamo di farci rappresentare da questo Governo nella stesura dei decreti delegati: non parteciperemo dunque alla votazione. Il suo Governo cambi metodo, apra un confronto serio e onesto su tutto, non solo episodicamente. Le diamo peraltro atto e diamo atto al relatore di aver avviato su questo provvedimento un confronto certamente costruttivo. Noi non ci tireremo indietro nel cercare di migliorare le vostre proposte, per fare leggi adeguate nell'interesse dell'Italia.

nasce da un *blitz* del Governo in sede di discussione di legge finanziaria, ce lo ricordiamo tutti. Un ordine del giorno voluto della maggioranza di questo Parlamento decise di bloccare quel *blitz* con un disegno di legge.

Ebbene, la maggioranza ha aderito ai nostri emendamenti votandoli. Ma cosa significa questo, Presidente? La maggioranza non era d'accordo con il disegno di legge delega presentato dal Governo.

perché, a detta di tutti ed anche di questa maggioranza, i nostri ricercatori sono i migliori al mondo: con le poche risorse sono quelli che producono di più; diamo loro maggiori finanziamenti. No! Ci si inventa e si gira intorno ai disegni di legge per parlare di ricerca, per porre al centro dell'attenzione la ricerca scientifica. Ma è un falso modo di porre l'attenzione della ricerca scientifica. Ebbene, mi dispiace che alcuni colleghi dell'opposizione votino diversamente dal resto della Casa delle Libertà. Mi dispiace per un doppio motivo: perché

o hanno sbagliato allora o sbagliano oggi! Votare una legge delega, comunque sia, da parte dell'opposizione, non significa altro che dare un voto di fiducia al Governo. Ebbene, dobbiamo prendere atto che alcuni hanno intenzione di dare il voto di fiducia a questo Governo. Ne prendiamo solamente atto. Noi, signor Presidente, non ci assentiamo. Ho molto apprezzato - perché no il relatore Ranieri quando ha consentito all'opposizione di porgli forti paletti alla legge delega iniziale, ma ho spiegato che non lo ha fatto per bontà, ma perché era intenzionato a farlo comunque, essendo nel suo interesse e della sua maggioranza porre dei paletti. È questo il problema. Pertanto il Gruppo Forza Italia, signor Presidente, non voterà e non parteciperà al voto. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tutti sappiamo come la situazione della ricerca in Italia appaia assai critica e tutti sappiamo come oggi si imponga un'azione costruttiva e al tempo stesso nuova, se vogliamo concretamente affrontare molte delle contraddizioni e delle inquietudini che la animano. Abbiamo davanti un'aritmetica certamente difficile, legata ad un numero di addetti per milione di abitanti nel campo della ricerca in Italia decisamente inferiore rispetto a quello degli altri Paesi europei e lo stesso rapporto con il prodotto interno lordo sviluppa livelli bassi, per molti versi discutibili. C'è però un dato in questo contesto che fa riflettere ulteriormente dalla produttività dei ricercatori italiani: una produttività che, al di là delle difficoltà, al di là dei limiti di natura economica, resta comunque alta, qualificata, autorevole. Noi valutiamo come ci sia il rischio di smarrire questa tendenza, di limitare i positivi riflessi che la ricerca in Italia anima e di azzerare in futuro la sua competitività. Arriviamo a questo provvedimento, come hanno sottolineato i colleghi, alla luce di un lungo approfondimento: un approfondimento critico che ha registrato il contributo utile e positivo di molti colleghi dell'opposizione e della maggioranza.

sviluppato un parere fortemente contrario al riordino degli enti di ricerca attraverso lo strumento regolamentare e voglio ricordare a tutti i colleghi che anche in Aula fu approvato un ordine del giorno che andava nella medesima direzione. Un pronunciamento preciso - e mi avvio alle conclusioni, signor Presidente - che ci ha spinti verso questo testo, considerando come ci siano obbiettivi dirimenti, fondamentali, che hanno caratterizzato il nostro lavoro: il coinvolgimento diretto della comunità scientifica nella delicata procedura di costituzione degli organi; il riconoscimento dell'autonomia statutaria degli enti; l'obiettivo raggiunto di abbandonare, finalmente, la zavorra della burocrazia nei singoli enti e di potenziare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori; l'opportunità di aderire ad un monitoraggio costante in questa fase transitoria. Si tratta di obiettivi concreti, sui quali si è animato il nostro lavoro e si è disegnata questa piattaforma comune, ricerca come fattore di sviluppo e come valore strategico da recuperare per il Paese. Ritengo che questo sia il valore di un'intesa che tende a riproporre il Parlamento al centro dei controlli e delle scelte decisionali del futuro. È sulla base di queste considerazioni che il Gruppo dell'Ulivo voterà a favore di questo provvedimento. Signor Presidente, innanzitutto desidero esprimere parole di ringraziamento al Sottosegretario Modica e al relatore Ranieri per l'attenta considerazione in cui hanno tenuto le mie

non è in relazione all'articolo 33 della Costituzione. L'autonomia statutaria è un'altra cosa. Sapete quale sarà la conclusione dell'autonomia statutaria? Sarà la seguente: una *governance* debole,

si tratta di una legge delega che mi vede contrario su tutta la linea e di cui non vedo le motivazioni. Soprattutto, essa non coglie i problemi veri e gravi della nostra ricerca, pertanto non porterà a nulla di buono.

Si tratta di dotare il Governo di strumenti rapidi per l'adempimento degli obblighi comunitari di attuazione di direttive. Tale provvedimento è molto richiesto dagli operatori finanziari per garantire la competitività in Europa ed Europa ed è necessario per evitare procedure di infrazione comunitaria. Mi appello dunque ai colleghi della maggioranza e dell'opposizione perché la discussione possa essere rapida e conclusiva.

Presidente, il Gruppo UDC non si è sottratto a un esame celere di un provvedimento che ridetermina i termini di delega per le direttive comunitarie in materia di autotrasporti, di OPA e di mercati degli strumenti finanziari, anche per i contenziosi comunitari in atto. Occorre però domandarsi perché siamo giunti a questo così grave ritardo

del fatto che la legge comunitaria n. 13, che all'articolo 10 conteneva il recepimento della direttiva, prevedendo anche modifiche alla legge n. n. 62, è stata pubblicata il 17 febbraio 2007, oltre un mese dopo l'approvazione parlamentare. Come si può vedere, Presidente, si tratta di un autentico groviglio legislativo che ha finito per determinare prima un grave infortunio, poi un autentico pasticcio, vanificando tutto il lavoro parlamentare. Forse il Ministro per le politiche comunitarie era troppo assorbito dalla funzione e dalle responsabilità del Dicastero per il commercio estero, per poter seguire una materia che richiede attenzione e partecipazione costanti. È lecito allora, da parte nostra, fare chiarezza rispetto a responsabilità che appartengono innanzitutto al Governo, perché il Parlamento ha fatto per intero la propria parte. Non può essere invocato l'alibi della contrapposizione: abbiamo voluto dare continuità alle nostre responsabilità di Governo nell'ambito della materia comunitaria. PRESIDENTE. è inutile che lei mi sollecita, perché ho alcune cose da dire. La ringrazio, non metta il turbo, perché noi vogliamo svolgere un ruolo di opposizione costruttiva! Ora con un emendamento della Commissione finanze la proroga viene ulteriormente differita al 30 settembre. Rispetto a tutto ciò, da parte nostra non abbiamo mai mancato di richiamare l'attenzione degli organi responsabili per intervenire prontamente. Lo stesso governatore Draghi, al Forex, ha sottolineato per il nostro Paese i riflessi derivanti da una maggiore concorrenza tra mercati regolamentati e le piattaforme gestite da grandi operatori, nonché la necessità per le banche di affrontare scelte decisive e tempestive. Dobbiamo dare atto alla Banca d'Italia di aver svolto un ruolo attivo e propositivo, di non essere rimasta inerte e, al Ministero dell'economia e delle finanze, di aver aperto un sito di consultazione con una relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, in attuazione delle deleghe previste dalla direttiva MIFID, proprio per guadagnare tempo. Non va dimenticato che su questa direttiva, definita da taluni un'autentica rivoluzione, si è registrato un alto livello di cooperazione istituzionale tra Parlamento Europeo, Commissione e Stati membri, un idoneo funzionamento della procedura Lamfalussy per conseguire un risultato adeguato per i mercati finanziari, per gli investitori e per i consumatori. rappresenta l'ultimo tassello, dopo le altre direttive sulla trasparenza, sul *market abuse* e sul prospetto, nell'integrazione dei mercati finanziari, realizzando un punto di equilibrio tra apertura ai mercati e principio della trasparenza. La rapida globalizzazione dei mercati finanziari è un'opportunità per l'Europa, perché possa diventare *leader*, se si guarda l'obiettivo di ridurre il costo del capitale, favorendo la crescita, migliorando le garanzie per gli investitori, migliorando la competitività nel suo complesso, così da aprire il mercato agli investitori. In sede europea sono emersi dubbi sulla flessibilità nel differimento della pubblicazione di informazioni sulle grandi operazioni e la interdipendenza delle operazioni inerenti agli strumenti derivati per non penalizzare i nuovi clienti e i nuovi mercati. Dobbiamo allora agire per un pronto recepimento della direttiva entro novembre, se vogliamo realizzare gli obiettivi, evitando i disallineamenti e le asimmetrie tra i mercati finanziari e borsistici nazionali. Le opportunità offerte dalla direttiva sono di gran lunga superiori alle sfide e la sfida sta nel costruire le piattaforme tecnologiche in grado di gestire le funzioni all'interno della piattaforma, perché si accresce la concorrenza, si migliorano i servizi, si riducono i costi per gli investitori, si favorisce l'apertura dei nuovi mercati, la possibilità per le società d'investimento di ripensare il *business,* di guadagnare in efficienza operativa e di centralizzare il *businness*. La MIFID ha imposto trasparenza *pre* e *post* *trade* solo per il mercato azionario, escludendo il mercato obbligazionario. Resta questa una questione aperta rispetto alle esigenze di maggiori informazioni, lasciando agli Stati membri un regime di trasparenza per gli strumenti finanziari diversi dalle azioni. Dobbiamo dare atto al ministro Bonino di avere espresso una chiara e distinta posizione, che apprezziamo, rispetto alla pesante azione del Governo sulla vicenda Telecom. Esprimiamo dunque preoccupazione perché il Governo non è stato neutrale, ma parte attiva, come dimostra la telefonata pubblicizzata da Bernheim del Ministro dell'economia allo stesso Presidente delle Assicurazioni Generali. Una regia occulta ha imposto una soluzione più politica che industriale, privilegiando un nocciolo finanziario espressione del cuore finanziario del Paese. Prevalgono i salotti buoni alle scelte di mercato. E infatti l'operazione è stata bocciata dal mercato, perché vi sono state troppe invasioni di campo. E il presidente Salza, presidente del consiglio di gestione di Intesa San Paolo, non è stato forse ricevuto il 2 aprile scorso a palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio? Troppi *rumors*? E non veniva forse questa visita collegata alla partita Telecom, allorquando si affermava che le banche non erano fuori dalla partita? E allora non abbiamo sentito riflessioni serie rispetto al tentativo di impedire un'operazione di mercato, prima quella con AT&T, che aveva carattere industriale più che finanziario, per poi ripiegare sulla subordinata telefonica, impedita a novembre perché portata avanti dall'azionista senza mediazioni della politica. Cosa c'entrano le assicurazioni con la telefonia? Quali sinergie industriali potranno mai generare? O forse è stata stipulata, com'è stato detto, una polizza assicurativa sul controllo delle Generali contro scalate interne? Non è forse il caso di far chiarezza? Il Presidente del Consiglio si è mosso come se fosse ancora il Presidente dell'IRI, con Mediobanca nel ruolo della finanziaria del gruppo telefonico, come se fosse ancora una partecipata delle BIN e con un una banca nel ruolo delle defunte tre BIN. Resta il giallo delle lettere alla CONSOB e resta il giallo dei comunicati. E, per stare al tema, che c'entrano gli investimenti delle banche nella telefonia, dichiarati strategici per i riflessi su Basilea 2, rispetto all'esigenza di investimenti nelle piattaforme tecnologiche e con gli obiettivi della direttiva MIFID? La vicenda Telecom è un pericoloso passo indietro rispetto all'esigenza di chiarezza e di trasparenza nell'affermazione di regole che esaltino la libertà economica piuttosto che controlli occulti, espressione non di un capitalismo democratico ma di qualcosa d'altro. Un'ultima considerazione: è stato detto che qualcuno considera Telecom come un'azienda di Stato. Ebbene: è sufficiente vedere gli *sponsor* televisivi della manifestazione di ieri del 1° maggio: in prima fila erano Telecom, del senatore Ciccanti)*. È questo il risultato di chi vuole una Telecom azienda di Stato. Il Gruppo UDC manifesta consenso sugli obiettivi della direttiva ma, al tempo stesso, non può rinunciare ad esprimere fortissime perplessità sul metodo seguito. Questo significa svolgere un'opposizione costruttiva, ma ferma rispetto agli errori compiuti dal Governo che hanno vanificato il precedente lavoro parlamentare e di cui chiediamo conto perché rappresenta un costo per il Paese.

permanente: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.100, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 2 venga aggiunto il seguente periodo: "Gli schemi dei decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE, sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni".